Onorevoli colleghi, nella seduta antimeridiana di ieri ho dato annunzio all'Assemblea della dolorosa scomparsa del collega senatore Luigi Scotti. Nato a Cernusco sul Naviglio il 19 gennaio del 1936, dopo brillanti studi classici (e di questa cultura classica andava meritatamente fiero, richiamandola spesso nel corso del suo impegno parlamentare, come ricorda chi ha avuto il piacere di frequentarlo da vicino), si era laureato in ingegneria, ottenendo, nel corso della sua lunga carriera professionale, delicati e prestigiosi incarichi di direzione aziendale. Dedicatosi più tardi, con grande passione, all'impegno politico, aveva saputo mettere al servizio della collettività la sua indiscussa levatura morale e le sue competenze tecniche ed organizzative. Divenuto membro di questa Assemblea nel 2001, era stato confermato dal corpo elettorale nelle due legislature successive. In questi sette anni di attività parlamentare, ci ha offerto una straordinaria testimonianza di dedizione al lavoro di senatore e grandissimo rispetto per l'Istituzione, rivelandosi tra i colleghi più assidui in assoluto nella partecipazione ai lavori dell'Assemblea e delle Commissioni parlamentari. Membro della Commissione ambiente, il suo impegno parlamentare sì è spesso concentrato sul tema attualissimo della gestione dei rifiuti, dimostrando su queste delicate questioni, ancor prima che le vicende campane le ponessero all'attenzione dell'opinione pubblica nazionale, una grande capacità di comprensione delle esigenze del tempo presente e di chiarezza nella priorità dell'azione dei pubblici poteri. A queste indubbie qualità politiche egli univa una grande ricchezza di doti umane: per il carattere solare, che faceva sì che dal suo volto non mancasse mai il sorriso, per la grande disponibilità ed attenzione che manifestava verso chiunque avesse a che fare con lui, Luigi Scotti era apprezzato e stimato da tutti i colleghi, che lo consideravano e lo apprezzavano come un vero galantuomo. La partecipazione alle sue esequie, che si sono tenute ieri pomeriggio a Cernusco sul Naviglio, mi ha consentito di percepire con commozione l'affetto, la stima e la grande considerazione di cui Luigi Scotti godeva all'interno della sua comunità e nel suo ambiente professionale. Voglio rinnovare ai suoi familiari, ed in particolare alla moglie Luciana - così duramente colpita dalla improvvisa ed inattesa scomparsa - e al figlio Davide, presente in tribuna, al quale indirizziamo un caro ed affettuoso saluto *(Generali applausi)*, la più sincera condivisione

più sincera condivisione del loro dolore, ed esprimere ai suoi elettori e ai colleghi del Gruppo parlamentare del Popolo della Libertà il cordoglio unanime della nostra Istituzione. Invito pertanto tutti colleghi ad osservare un minuto di raccoglimento.

prendere la parola per rendere l'ultimo saluto ad un collega e amico è sempre una situazione di estremo disagio. Sono situazioni che non si vorrebbero mai affrontare. Frequentando il senatore Luigi Scotti dalla XV legislatura, il ricordo più vivo che mi rimane in memoria è la sua vitalità, la bontà, le maniere semplici e la sua attenzione per le problematiche della società civile; infine, la sua disponibilità, il rispetto nei confronti dei colleghi e la sua apertura mentale anche per le ragioni di un avversario politico. Per concludere, posso solo dire che la sua sarà un'assenza che impoverisce umanamente e politicamente questa Assemblea.

onorevoli colleghi, siamo rimasti profondamente colpiti e addolorati dall'improvvisa scomparsa del senatore Luigi Scotti, di cui si ricorda l'impegno nel lavoro parlamentare nei suoi sette anni e mezzo a Palazzo Madama, con una presenza assidua in Aula e in Commissione. Lombardo, nativo di Cernusco sul Naviglio, ingegnere e dirigente aziendale in pensione, il senatore Scotti è stato eletto per la prima volta in Senato nel 2001. Durante le sue tre legislature consecutive si è fatto conoscere in tutta la sua semplicità e schiettezza, nella sua umanità, nonché nell'attenzione alle tematiche ambientali nel ruolo di membro della Commissione ambiente. Alla sua famiglia e al Popolo della Libertà va il più profondo cordoglio del Gruppo dell'Italia dei Valori per la perdita di un uomo onesto, molto attaccato alla famiglia e alla moglie Luciana, che andava a trovare - mi hanno detto i senatori lombardi suoi amici - tra una seduta e l'altra, spesso viaggiando anche di notte, per presenziare di buon mattino all'apertura dei lavori. Era un cattolico, impegnato nel sociale e nel volontariato. Aiutava i deboli e gli ultimi. Quindi, a Luigi Scotti, che credeva nei valori della famiglia, negli ideali e nell'impegno politico, da parte dell'Italia dei Valori, che la terra gli sia lieve*.

è difficile prendere la parola quando un amico ci lascia così improvvisamente, ma non posso

io avuto una formazione tecnica e non classica. Così, con l'inizio di questa legislatura, avevamo fatto

sovrintendeva il tutto la senatrice Mazzuconi, che latino invece lo insegna sul serio, e ci metteva poi alla prova.

per approfondire le lezioni di latino. Il suo carattere razionalista, da ingegnere, andava a scontrarsi un po' con il mio carattere eclettico di architetto: a lui, così razionale, piaceva il calcio, a me il ciclismo; lui da giovane era amante della Lambretta, io ho sempre avuto la Vespa. Ma proprio questa differenza, che poi è quel filo del federalismo che unisce nelle diversità,

sono andato a cercare due frasi in latino, per fare onore alla sua cultura latinista, alla sua memoria: «*Venit mors velociter, rapit nos atrociter, nemini parcetur. Nos habebit humus»*, vale a dire: «La morte viene velocemente, ci rapisce atrocemente, nessuno sarà risparmiato. La terra ci possiederà».

Non è agevole, in generale, parlare in modo sensato delle persone che si incontrano e con le quali si condivide un'attività e un impegno per un tratto non lungo. In questo caso il mio compito è ancora più difficile perché in quest'Aula sono presenti colleghi che con il senatore Scotti hanno condiviso addirittura l'esperienza sui banchi di scuola, fin dai primi studi, e che a lui, dunque, sono legati da consuetudine antica e robusta. Cercherò tuttavia, con rispetto e attenzione, di intervenire su ciò che ho visto e ho capito di lui, uomo aperto e schietto, senza infingimenti e con non comuni doti umane.

Questa sua attitudine è andata ben al di là dei comuni e talvolta freddi rapporti di pura cortesia. Indagatore attento di fatti e persone, comunicava serenità e amore appassionato alla vita. Uomo di fini conoscenze umanistiche, come ben si costumava agli ingegneri lombardi di un tempo e di un mondo forse perduto, e di cui la terra lombarda annovera insigni esempi, egli non trovava tra la sua formazione tecnica e le radici classiche della sua cultura alcuna frattura, bensì continuità e logica connessione. Ne ho apprezzato la piacevole conversazione e l'attitudine giocosa e insieme seria nell'utilizzo della lingua latina, che egli amava e che ricordava volentieri, come volentieri rammentava il tempo trascorso nelle aule della scuola salesiana, che aveva frequentato in anni lontani. Proprio da quella scuola, oltre che dall'indole naturale, aveva probabilmente riportato il suo positivo atteggiamento verso la vita, il lavoro e le persone. Nonostante fosse pervenuto in anni abbastanza recenti alla politica non l'ho mai sentito dire di essere un uomo "prestato alla politica", come si suol dire oggi in un modo snobistico e vagamente dispregiativo, che nega alla politica il ruolo e il valore che la contraddistinguono, quando essa non viene assolutizzata e non schiaccia le persone. Luigi Scotti non era snob, né tantomeno aveva un atteggiamento negativo sull'esperienza della vita e in particolare sulla politica in questa fase della sua vita, anzi. vita, anzi. Luigi Scotti, come peraltro è stato detto ieri ai suoi funerali, era uomo semplice e tutto d'un pezzo, politico franco e vicino alla gente, per la quale contavano e contano i problemi quotidiani da risolvere e non un dibattito altisonante e sterile, magari amplificato dalla comunicazione mediatica. Il senatore Scotti di questo è stato consapevole e attivo testimone. Democratico vorrei dunque ricordare il senatore Luigi Scotti, pur nella diversità delle opzioni politiche, come uomo degno di stima e di onore, come un uomo che ha preso molto sul serio la famiglia e il lavoro e si è dedicato ai problemi quotidiani della gente. Vorrei ricordarlo anche come collega preparato e dialogante, appassionato alle questioni che ci vengono affidate nel lavoro quotidiano in Senato, ma soprattutto come uomo vero, come uomo buono, capace di un confronto leale e di relazioni umane profonde e attente all'altro, qualunque opinione esprimesse o rappresentasse. Ricordiamolo dunque così: uomo di dialogo, fermo nelle sue convinzioni e soprattutto ricordiamone il sorriso, indice certo che le persone e il mondo circostante non gli erano mai indifferenti.

Signor Presidente, mi accingo con commozione a ricordare brevemente l'amico carissimo, senatore Luigi Scotti, improvvisamente scomparso nel sonno, a casa sua, sabato scorso 6 dicembre. Una morte totalmente inaspettata che ha lasciato per questo ancora più costernati, affranti e sgomenti prima di tutto i familiari, ma duramente colpiti anche tutti noi che lo conoscevamo e gli volevamo bene. Luigi, a quasi 73 anni, era nel pieno delle sue forze: fisico asciutto e robusto (da giovane era stato un ottimo giocatore di calcio), controllava da anni, senza sgarrare, la propria alimentazione e faceva regolare esercizio fisico. Mai una malattia. Tutto bene anche nell'ultimo *check up* periodico, eseguito qualche giorno fa. Purtroppo, però, la morte arriva lo stesso. Era nato il 19 gennaio 1936 a Cernusco sul Naviglio, una cittadina a una decina di chilometri da Milano, che amava molto, in cui avrebbe abitato gran parte della sua vita, in cui avrebbe concluso i suoi giorni terreni. La sua famiglia di origine, economicamente assai modesta, era una di quelle sane famiglie di una volta, ben radicate nel territorio, con un accogliente parentado di nonni, zie e zii, cugine e cugini. Il padre operaio meccanico all'Alfa Romeo, la madre sarta, un fratello minore, Vito. Una vita familiare ricca di valori preziosi: spirito di sacrificio, industriosità, solidarietà, serenità degli affetti. Intelligenza viva e rapida, serio, studioso, memoria di ferro, Luigi si fa subito notare come ottimo scolaro alle elementari. Nel 1947 i suoi affrontano di buon grado il sacrificio di mandarlo come interno alla scuola media dei Padri salesiani dell'istituto Sant'Ambrogio di via Copernico a Milano. Riesce molto bene, primo della classe in tutte e tre le medie. Passa poi al ginnasio, al liceo classico, sempre nello stesso istituto, sempre con ottimo successo negli studi, appassionandosi in particolare al latino, al greco e all'italiano, come è stato ricordato prima. Ancora a 70 anni si districa benissimo con il latino e ricorda a memoria centinaia di versi di poesie di Leopardi, di Foscolo, di Manzoni. Diploma di maturità classica nel luglio del 1955. Nella sua classe, al ginnasio e al liceo, una classe rimasta molta unita in tutti questi anni, c'era anche Silvio Berlusconi che ovviamente ha avuto modo di conoscerlo a fondo, di stimarlo e di divenirne amico. In quella classe abbiamo avuto la fortuna di esserci anche il senatore Romano Comincioli ed io. Nell'ottobre 1955 si iscrive alla facoltà di ingegneria industriale (elettrotecnica) del Politecnico dì Milano, università allora particolarmente severa, che termina all'inizio del 1963. Appena laureato viene subito assunto dalla SIP (ora Telecom Italia). Compie presso questa grande società l'intera sua carriera di lavoro, fino alla pensione nel 1995. Sono i decenni del rapido sviluppo della rete telefonica fissa, fondamentale infrastruttura del nostro Paese. In azienda si accorgono subito delle doti del neoassunto: affidabilità, dedizione, capacità di guida delle persone, competenza tecnica, concretezza, ottima capacità relazionale. Gli vengono affidate responsabilità via via crescenti: impiegato, quadro, dirigente, infine direttore di distretto telefonico, con grosse responsabilità gestionali e manageriali in varie sedi di lavoro: Cremona, Brescia, Monza, infine Milano in via Washington. Si sposa il 7 giugno 1969 con la signora Luciana Andretta, professoressa di lettere nella scuola media, che continuerà ad insegnare fino al momento della pensione. Il matrimonio è presto allietato dalla nascita di un figlio, Davide (nel marzo 1970). Alla famiglia Luigi ha dedicato sempre appassionata attenzione, rispondendo con grande sensibilità alle esigenze derivanti dai tanti ruoli ricoperti: figlio, fratello, marito, padre, suocero, nonno (di due splendide nipotine). Dopo l'entrata in pensione, libero da impegni di lavoro, inizia nel 1996 ad occuparsi attivamente di politica. Collabora con chi vi parla nell'azione di coordinamento dei club Forza Italia, sorti in pochissimo tempo a migliaia nel 1994 con la discesa in campo di Silvio Berlusconi. Contribuisce con il suo buon senso e la sua misura alla delicata azione di incanalamento di queste impetuose e vigorose energie della società civile nella struttura ordinata di un grande partito liberale di massa, Forza Italia, allora in costruzione. Nel 1997 il sindaco di Milano Gabriele Albertini lo nomina membro del consiglio di amministrazione della società AMSA, la società che cura la raccolta e la gestione dei rifiuti solidi urbani della città di Milano. È qualificato per questo importante incarico per merito della sua esperienza manageriale. Farà fronte a tale impegno con generale apprezzamento e l'incarico gli verrà così rinnovato più volte fino al 2007. Nelle elezioni politiche del 2001, candidato della Casa delle Libertà nel collegio senatoriale n. 15 di Melzo nella circoscrizione della Lombardia, viene eletto senatore per la prima volta. Per questa XIV legislatura sceglie di inserirsi nella Commissione ambiente, dove ha modo di far valere la sua esperienza nel settore dei rifiuti acquisita nel consiglio d'amministrazione dell'AMSA. Inoltre, nella stessa legislatura è membro della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, nonché del Comitato parlamentare per i procedimenti di accusa. Si distingue, tra l'altro, per la grande assiduità della presenza parlamentare. Viene eletto senatore una seconda volta nell'aprile 2006, sempre in Lombardia, nelle file di Forza Italia. In questa XV legislatura è di nuovo membro della 13a Commissione permanente ed altresì membro della Commissione consultiva per la concessione delle ricompense al valore e al merito civile. Al Senato, data l'esigua differenza numerica di voti esistente tra lo schieramento della maggioranza di centrosinistra e il centrodestra (appena tre voti), lo scontro tra maggioranza ed opposizione è molto combattuto. In particolare, diventa di estrema importanza la compatta presenza al voto in Aula. Il senatore Scotti contribuisce sempre con il massimo impegno a questa così rilevante azione di militanza politica. È eletto senatore una terza volta nelle elezioni del 13 e 14 aprile di quest'anno, sempre in Lombardia, nelle file del Popolo della Libertà. Anche in questa legislatura è membro della 13a Commissione permanente. Cattolico praticante, Luigi Scotti si è sempre ispirato nella sua vita ai valori cristiani trasmessigli dalla famiglia e dall'insegnamento dei padri salesiani. Cari colleghi, perdiamo con il senatore Luigi Scotti una persona rara, profondamente buona, integerrima, generosa, rispettosa degli altri, sempre disponibile, affidabile, leale e con un alto senso del dovere. Sono tutte virtù umili, poco appariscenti, ma così importanti anche in politica. Luigi è stato un fulgido esempio della validità della scelta per la rappresentanza parlamentare anche di persone provenienti dalla vita civile, che in essa abbiano dato ottima prova delle proprie capacità. Nei suoi interventi qui al Senato abbiamo tutti potuto apprezzare il suo buon senso, la visione equilibrata dei problemi, il sano realismo, la cultura del "fare" propria dell'ingegnere, la profonda conoscenza degli uomini, frutto dell'esperienza manageriale. Al funerale di ieri, a cui tanti colleghi, loro malgrado, non hanno potuto essere presenti per le inderogabili esigenze della vita parlamentare, vi è stata un'amplissima partecipazione della comunità dei cittadini di Cernusco. Chi è stato alla toccante cerimonia ha potuto constatare quanto le virtù semplici e miti di Luigi, la sua vita tra la gente, la sua cordiale disponibilità siano state sentite ed apprezzate dai cittadini come un modo nuovo ed esemplare di vivere l'impegno politico. Addio, carissimo Luigi! Ci mancherai tanto! In questo commiato, vorrei ricordare alcuni versi di una poesia che ti era cara: «Non vive ei forse anche sotterra, quando gli sarà muta l'armonia del giorno, se può destarla con soavi cure nella mente de' suoi? Celeste è questa corrispondenza d'amorosi sensi, celeste dote è negli umani; e spesso per lei si vive con l'amico estinto e l'estinto con noi...».

Onorevolicolleghi, ho ricevuto oggi dal Capo dello Stato la seguente lettera a me indirizzata, di cui do volentieri lettura all'Assemblea: «In occasione della ricorrenza del Sessantesimo anniversario della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, desidero unirmi a quanti sono impegnati, in Italia e nel mondo, per affermare e garantire il primato della persona e della sua dignità su basi di libertà e di eguaglianza. In tale azione trovo ispirazione nei principi nella nostra Carta costituzionale, di cui abbiamo celebrato quest'anno i sessant'anni anni di vita, e che vengono riaffermati nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo e nei Trattati istitutivi dell'Unione europea. La Dichiarazione del 1948 ha affermato il valore essenziale della dignità umana, ovunque nel mondo, senza distinzione di razza, sesso, lingua, religione o opinione, cittadinanza o *status* sociale. Adottando quel documento, la Comunità internazionale ha riconosciuto che il primato dei diritti della persona è condizione basilare per realizzare concretamente la pace, la libertà e la giustizia tra i popoli. I principi sanciti nella Dichiarazione sono stati progressivamente oggetto di numerose convenzioni internazionali, che hanno dato vita ad un vasto patrimonio normativo. Tale processo evolutivo, particolarmente rilevante e fecondo in ambito europeo, ha rafforzato la consapevolezza della responsabilità internazionale per la tutela dei diritti umani e della necessità di prevedere adeguati sistemi di verifica da parte degli Stati. Ciò nonostante, dobbiamo purtroppo constatare il profondo divario che ancora oggi separa le enunciazioni dei diritti dal loro effettivo esercizio. Mentre in tante parti del mondo antiche violazioni non sono scomparse, la tutela dei diritti deve infatti affrontare nuove minacce legate al terrorismo, alla tutela dell'ambiente ed ai cambiamenti climatici, alle lesioni della *privacy*, all'impatto delle crisi economiche sulla condizioni di vita dei singoli e delle collettività. La doverosa constatazione dell'insufficienza degli sforzi sinora compiuti impone un rinnovato e più forte impegno da parte delle istituzioni, delle associazioni e dei singoli per prevenire ogni ingiustificata violazione dei diritti e garantirne la loro tutela. Il Parlamento può dare certamente un impulso cruciale in tale direzione. Mi auguro, infine, che la celebrazione odierna contribuisca ad avvicinare sempre più i nostri giovani al contenuto della Dichiarazione, aiutandoli a coltivare il senso profondo di una fratellanza basata su principi e valori universali, che essi dovranno saper condividere, trasmettere e difendere ovunque nel mondo. *F.to* Giorgio Napolitano».

e nel giorno del 60° anniversario della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, che proprio oggi, per iniziativa del Gruppo interparlamentare «Amici della Birmania», la stessa cosa avviene alla Camera per iniziativa della collega Margherita Boniver) una mozione per richiamare l'attenzione del Parlamento, del Governo, dell'intera Unione europea e del consesso internazionale sui diritti violati in Birmania. affinché il popolo birmano e Aung San Suu Kyi sappiano che i popoli e le istituzioni democratiche del mondo che amano la libertà sono con loro. Spero poi che quanto prima sarà possibile discutere la mozione nella nostra Aula. *(Applausi

questa mattina un normale cittadino che avesse ascoltato o letto il contenuto dell'emendamento 1.0.1-*bis*, presentato dal Partito Democratico, e poi avesse ascoltato il parere negativo su quell'emendamento, con le sue motivazioni, del sottosegretario Vegas avrebbe potuto avere percezione chiara dell'alternativa di politica fiscale e di bilancio che in questo momento viene presentata dal Governo in carica e dal principale partito di opposizione. In sostanza, il sottosegretario Vegas, di fronte ai contenuti della nostra proposta,

questione di sede: la sede dentro cui collocate queste proposte per il Governo è inappropriata; il Governo considera sede appropriata il decreto n.

di segno della politica di bilancio del Governo, di segno della politica di bilancio proposta dal Partito Democratico ed è di segno perché, in buona sostanza, il Governo ci dice che non intende modificare il segno il Partito Democratico propone un mutamento netto di segno, da restrittiva ad espansiva, della politica di bilancio per il 2009, con la garanzia - ho già spiegato attraverso quali proposte - che nel 2010, 2011 e 2012 vi siano gli effetti di misure da approvare immediatamente, che siano in grado di ridurre la spesa corrente primaria, facendo così ritornare la finanza pubblica in un alveo di stabilità.

ma ciò che differenzia le soluzioni qui contenute, a causa della cornice di cui ho detto, rispetto alle proposte contenute nel decreto n. 185, è che quel decreto non può contare su un volume di risorse adeguato (un punto di prodotto interno lordo) per fare delle misure che contiene non semplicemente delle inutili e inefficaci allusioni a delle politiche di contrasto della crisi e della recessione in atto, ma degli interventi che abbiano effettività e capacità di incidere. La differenza è questa e non sarà il titolo delle misure, ma il loro carattere economico a fare la differenza.

Presidente, onorevoli colleghi, il Gruppo del Partito democratico in 9a Commissione si è fatto carico di una serie di emendamenti, volti a stabilire adeguati sostegni a due settori in crisi come l'agricoltura e la pesca così da promuoverne il rilancio. Confido naturalmente nell'accoglimento degli stessi, insieme con i miei colleghi, e mi limito ad illustrarne uno soltanto, il 2.1, relativo ad un incremento del Fondo di solidarietà nazionale per di solidarietà nazionale per 200 milioni di euro - questa è la nostra proposta - per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, al fine di dare piena attuazione ai meccanismi di gestione del rischio in agricoltura e di potenziare il ruolo delle polizze assicurative. Con la legge 29 novembre 2007, n. 222, di conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, recante interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale, collegato alla finanziaria 2008, la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale per le calamità naturali (interventi assicurativi) è stata incrementata di 30 milioni di euro per integrare il contributo alle imprese agricole nel 2007 ed ed arrivare a 220 milioni di euro, visto che con la legge finanziaria del 2007 erano stati stanziati 190 milioni di euro. Uno strumento, quello del Fondo di solidarietà nazionale, di importanza vitale per contenere i rischi che si paventano in qualsiasi attività agricola, attraverso il quale i produttori possono stipulare polizze in forma collettiva aderendo ad uno dei consorzi di difesa oppure ad una cooperativa che esercita l'attività di difesa a favore degli associati.

Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, proprio considerando l'importanza strategica della risorsa idrica per la qualificazione del settore agricolo e per promuovere un'agricoltura di precisione sono necessari interventi che possano garantire il risparmio idrico e, soprattutto, una corretta gestione delle acque. A tale riguardo, le finanziarie varate dal precedente Governo avevano dato priorità al concreto e fattivo rilancio degli investimenti del piano irriguo nazionale ed anche all'ottimale gestione delle risorse allocate, pari a 100 milioni di euro per l'esercizio 2007 ed a 150 milioni di euro per gli esercizi 2008 e 2009. Venendo ad oggi, tanto il decreto n. 112 quanto la finanziaria 2009 non hanno previsto al loro interno specifiche misure per la risoluzione dell'emergenza idrica in agricoltura, né per il rilancio del piano irriguo nazionale. Anzi, la finanziaria 2009 ha previsto un taglio pari a 50 milioni di euro per gli investimenti sul piano irriguo nazionale. tale scopo, l'emendamento 2.2 vuole stanziare risorse finanziarie pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009-2011. Crediamo che soltanto attraverso questo tipo di intervento si potrà davvero garantire l'avvio ed il completamento delle opere previste nel piano irriguo nazionale, nel tentativo di fornire possibili soluzioni all'emergenza idrica in Basilicata e di dare risposte certe agli operatori del settore. un'emergenza idrica che stanno vivendo in questo momento le regioni Puglia e Basilicata e che non penalizza soltanto il settore agricolo, ma che mette a rischio tanto il settore civile quanto quello industriale.

ispettivo in merito al riconoscimento della crisi idrica in Basilicata, assegnando un contributo straordinario per la realizzazione delle opere irrigue ritenute urgenti e prioritarie.

prevede agevolazioni per le imprese agricole in aree svantaggiate, quindi Mezzogiorno e montagna, in merito ai contributi previdenziali. Voglio ricordare che è stato introdotta, con emendamento approvato in quest'Aula al decreto-legge n. 171 del 2008 in materia di competitività del sistema agroalimentare, una proroga di dette agevolazioni al 31 marzo

costituiscono la disponibilità finanziaria per questo rinvio al 31 marzo 2009 sono stati sottratti da importanti provvedimenti a favore del settore agricolo-alimentare; mi riferisco sia al credito d'imposta per i certificati di controllo di qualità

di 459 milioni di euro gli stanziamenti previsti per il Ministero delle politiche agricole - è evidente che ulteriori tagli per riuscire a coprire

Presidente, colleghi, intervengo a sostegno dell'emendamento 2.6 riguardante l'imprenditoria giovanile femminile. È di qualche ora fa la dichiarazione del ministro Zaia

adotteranno strumenti per consentire il loro ingresso. La stessa cosa emergeva dal rapporto Nomisma di qualche giorno fa sulla competitività dell'agricoltura italiana, cui si evidenziavano ritardi strutturali. Da un lato, la polverizzazione aziendale e la frammentazione poderale, che non consentono di sfruttare al meglio tecnologia ed innovazione e quindi di realizzare la cosiddetta filiera corta, dall'altro la senilizzazione della nostra agricoltura,

Signor Presidente, intervengo per illustrare gli emendamenti 2.8 e 2.15. Si tratta di due emendamenti che intendono riaffermare due principi valoriali che interessano trasversalmente la maggioranza e l'opposizione. Sono principi generali, accettando l'indicazione del

Tremonti, il quale si è dichiarato non a conoscenza di questo elemento. Se prima potevamo accettare l'elemento di non conoscenza, oggi pensiamo che debba essere dato un giudizio di merito, sia da parte dei relatori che da parte del Governo, rispetto alla

emendamenti a cui intendo riferirmi direttamente, espressione di un lavoro svolto dai componenti del Gruppo del Partito Democratico in 6ª Commissione, vorrei evidenziare tre aspetti. di essi è quello che si esplicita principalmente negli emendamenti 2.14, 2.16 e 2.450, tutti tesi a ribadire la necessità di rispondere alle difficoltà economiche di tante famiglie e di favorire, in uno spirito di equità sociale, il recupero di un po' di potere di acquisto per diverse tipologie e categorie di persone. Va in questa direzione - lo voglio sottolineare - l'adeguamento l'adeguamento cui ha fatto riferimento il collega Musi e che tarda ormai da 13 anni, della misura che definisce la soglia di reddito al di sotto della quale i familiari si considerano a carico e che oggi è parametrata su 2.840,51 euro.

Dunque, all'esiguità della tutela si aggiunge la beffa: più le persone sono meritevoli e più vengono penalizzate. Ancora, proponiamo di intervenire sulle sofferenze delle famiglie che hanno subito l'aumento dei mutui per per l'acquisto della prima casa innalzando la quota detraibile. Proponiamo inoltre di intervenire con misure di alleggerimento della pressione fiscale sui redditi dei pensionati, con la costituzione di un fondo *ad hoc*, che è altra cosa e, se mi si consente, è migliore cosa della *social card*. Tralascio ogni valutazione circa l'aspetto caritatevole di quest'ultimo intervento, ma vorrei soprattutto evidenziare che lo strumento è macchinoso, inadeguato e di limitatissimo impatto. Il secondo punto che intendo evidenziare riguarda misure di semplificazione nel rapporto con gli intermediari e i contribuenti di lavoro autonomo e di piccola impresa, l'esigenza di potenziare l'azione di controllo e contrasto all'evasione ed elusione fiscale con un'attenzione particolare alla dotazione di mezzi e risorse per la Guardia di finanza, e una ricerca di innovazione con l'introduzione di una sperimentazione per modalità che consentano di velocizzare i pagamenti tra pubbliche amministrazioni e loro fornitori, consentendo la compensazione dei crediti per una somma fino a 10.000 euro una volta decorso un tempo congruo riconosciuto per il pagamento. Il terzo punto riguarda invece la questione degli emendamenti che puntano a sostenere gli investimenti. Si tratta di un altro tema importantissimo su cui abbiamo insistito e continueremo ad insistere nel corso della discussione, perché diversi di questi emendamenti riprendono un tema già illustrato dal collega Stradiotto, circa le modifiche al Patto di stabilità per liberare risorse che gli enti locali potrebbero orientare in direzione di opere accantierabili velocemente e in grado di apportare dinamismo alle economie dei rispettivi territori. Infine, vorrei sottolineare un aspetto a cui teniamo molto come Partito Democratico: l'uso della fiscalità in funzione di sollecitazione di interventi che stimolino l'emersione di gettito e siano motore per l'incentivazione di nuove opportunità di lavoro, con modalità che valorizzino la convergenza di interessi tra imprese, fornitori e contribuenti. Mi riferisco, in particolare, all'emendamento 2.173, che tende ad allargare la filiera dei meccanismi di agevolazione sulla norma che premia con il 36 per cento di sgravi fiscali le ristrutturazioni edilizie. Sottolineo il senso della norma, che va in direzione opposta alle restrizioni introdotte con il decreto n. 185 sulle misure di risparmio energetico. Soprattutto, vorrei mettere in evidenza il suo valore in funzione di trasparenza e di deterrenza verso i rischi di opacità, che in un settore in un settore come quello dell'edilizia potrebbero invece venire accentuati in questa fase di difficile momento economico e quindi di difficoltà sia per le imprese che per le famiglie. Mi auguro che chi si dice così attento al tema della sicurezza non guardi solo alla propaganda, ma sia disponibile ad agire di conseguenza e in un'ottica di prevenzione dei rischi, oltre che nell'interesse dell'erario.

prevede - qualora venisse approvato - il riconoscimento in termini effettivi e stabili alla detraibilità degli oneri per carichi di famiglia anche ai cittadini italiani non residenti sul territorio nazionale

al fine di dare un importante segnale ai numerosi connazionali residenti all'estero che attendono il riconoscimento di tale diritto, nonché per assicurare tutti i cittadini italiani, indipendentemente dalla loro residenza, analogo trattamento tributario.

L'emendamento 2.202 mira a colmare un'ingiustizia conseguente ad un vuoto legislativo: la legge n. 448 del 2001 prevedeva la possibilità per l'acquirente di un'unità immobiliare, facente parte di un fabbricato oggetto di restauro o ristrutturazione edilizia, di detrarre dall'IRPEF parte del valore degli interventi eseguiti. Queste detrazioni sono state negli anni prorogate, tranne però che per gli interventi di ristrutturazione avvenuti nel 2007. Ossia, se la compravendita riguarda un immobile facente parte di un edificio ristrutturato nel 2007 e solo in questo anno, l'acquirente non ha diritto di beneficiare della prevista detrazione. Con l'emendamento2.240 si propone l'incremento dell'importo della pensione spettante ai ciechi totali e ai ciechi parziali.

dei contratti dei pubblici dipendenti contrattualizzati, mentre il 2.252 riguarda la somma destinata ai miglioramenti economici del rimanente personale statale in regime di diritto pubblico. Proseguendo

che la sede per la determinazione dei trattamenti accessori per i pubblici dipendenti è la contrattazione integrativa. si ribadisce che la sede per la determinazione dei trattamenti accessori per i pubblici dipendenti è la contrattazione con le organizzazioni sindacali più rappresentative. L'emendamento 2.289 prevede che può essere altresì devoluta al finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni una quota parte delle risorse eventualmente derivanti dai risparmi aggiuntivi.

all'incremento del Fondo per interventi straordinari di edilizia scolastica. In tema di riduzione dei costi della politica,

elimina la cumulabilità dell'indennità da Ministro con quella da parlamentare. Si parla tanto di "casta" eppure, quando bisogna votare questi emendamenti

(l'abrogazione dei suddetti commi riporterebbe l'organico degli insegnanti di sostegno al livello dell'anno scolastico 2007-2008), mentre l'emendamento 2.0.57 consente anche ai presidi che nell'anno scolastico 2006-2007 risultavano destinatari di incarico di presidenza, nelle more di svolgimento delle prove concorsuali,

Con questo emendamento intendiamo sottolineare che tale disposizione, nel caso di aziende costrette ad una poderosa esposizione finanziaria per completare il ciclo di produzione di tali prodotti, comporta irrimediabilmente

purtroppo ormai di entità modestissima - proprio per favorire le lunghe stagionature. Ricordo che giornalmente le aziende socie di consorzi di tutela comprano la materia prima, pagando entro i primi 60 giorni

del TUIR tutte le aziende che non possono fare a meno di stagionare il prodotto alimentare per molti mesi e che si vedono costrette ad importanti approvvigionamenti finanziari per l'ineluttabile gestione del magazzino.

I Comuni italiani non sono mai stati in difficoltà come in questo periodo: da una parte c'è il taglio dei trasferimenti, dall'altra il mancato riconoscimento del 100 per cento dell' ICI come mancato introito. L'altra questione importante da considerare è la forte contrazione delle entrate proprie derivanti dagli oneri di urbanizzazione: il crollo del mercato immobiliare ha fatto sì che in questi mesi si assista al crollo delle entrate proprie, perché gli oneri di urbanizzazione non entrano più nelle casse dei Comuni. A questa situazione difficile si aggiunge il Patto di stabilità che impedisce di fatto, soprattutto agli enti più virtuosi, di

il nostro Gruppo ha presentato una serie di emendamenti che, in sintesi, si concentrano su due forti richieste

il secondo punto su cui convergono una serie di emendamenti è l'alleggerimento dei pesi burocratici per le imprese, soprattutto per quelle piccole e medie. - prevedeva una proroga dei termini per il libro unico del lavoro che ci sembrava sensata per poter meglio organizzare

significa che si mette a rischio il sistema pensionistico, ma anche tutto il sistema sociale, perché una fascia sempre più esigua di giovani deve mantenere una fascia crescente di persone anziane.

o servizi utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti volontariamente sostenute per finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto.

a carico delle aziende in forme diversificate e molto complicate, perché i dipendenti possono essere iscritti a vari fondi pensione con modalità diverse. Ancora sul settore pensionistico, è previsto finora che i coltivatori diretti possano scegliere una fascia superiore per i loro contributi e la relativa pensione. Con l'emendamento

vorremmo ampliare il termine per le comunicazioni di assunzione di lavoratori. È previsto dalla nuova legislazione che il rapporto di lavoro deve essere comunicato il giorno antecedente all'inizio del rapporto di lavoro: ci sembra poco realistico e impossibile, soprattutto in certi settori come ad esempio il turismo

potrebbe aiutare l'Italia ad affrontare il problema dell'equiparazione dell'età pensionabile tra uomo e donna. Seguiamo quest'obbligo europeo, ma aiutiamo le donne prevedendo per ogni figlio che hanno partorito o comunque educato, anche adottato, un periodo da detrarre

sul tema degli asili nido. L'Italia è in gravissimo ritardo da questo punto di vista, ma la nostra non è solo una scelta di carattere culturale, è una scelta di carattere familiare ed economico che si inserisce nelle scelte richieste dall'Unione europea,

un numero di asili nido che coprano almeno il 33 per cento del fabbisogno nazionale. Noi oggi ci attestiamo sul 6 per cento, con una disparità territoriale abissale: una minore presenza in Regioni soprattutto del Centro-Sud, in modo particolare del Sud, rispetto a quelle del Nord; Regioni come l'Emilia-Romagna e la Lombardia hanno un'offerta in numero di asili nido

agli altri Paesi europei, non i Paesi che sono entrati da pochi anni, ma quelli che storicamente, con noi, hanno costituito l'Europa.

Io non sono legatissima ai numeri e ai dati, ma questi ho voluto presentarli per mettere in evidenza l'abisso Invito quindi il sottosegretario Vegas, il Ministro e anche la maggioranza dei parlamentari, sia del Popolo della Libertà che della Lega a considerare con attenzione questi emendamenti perché essi vanno nell'ottica di coprire una richiesta proveniente dalla famiglia. Non possiamo sostenere la famiglia solo a livello ideale: tutti ci riempiamo la bocca ma poi concretamente non facciamo nulla. vanno anche nell'ottica di favorire una maggiore occupazione femminile, che rappresenta un altro buco nero del Paese Italia. Noi abbiamo il tasso di occupazione femminile più basso in Europa rispetto al confronto con gli altri Paesi europei.

non comprendo. Ho presentato molti altri emendamenti e mi riservo di intervenire per illustrarli quando saranno posti in votazione. Intervengo adesso su un aspetto riguardante la dichiarazione di inammissibilità degli emendamenti a mia firma, 2.132, 2.133 e 2.142, dichiarati inammissibili perché ritenuti localistici dalla Commissione. Tale dichiarazione contraddice il testo normativo perché questi emendamenti riguardano

che riguarda specificatamente misure per favorire la ricostruzione e la riparazione di immobili distrutti o danneggiati nei Comuni della Valle del Belice colpiti dal terremoto, è una norma sostanziale del il presunto carattere localistico dei miei emendamenti è comune sia alla norma del testo governativo che agli emendamenti. Non essendo stata segnalata dal Presidente del Senato in fase preliminare alcuna incompatibilità della norma dell'articolo 2, comma 9, con le regole della legge di contabilità, ne consegue che va considerata ammissibile ogni modifica o integrazione di tale disposizione con emendamenti, anche aggiuntivi.

Quindi, chiedo alla Presidenza di riconsiderare l'inammissibilità e di ammettere alla discussione e alla votazione gli emendamenti a mia firma, cioè il 2.132, il 2.133 e il 2.142, perché vi è una evidente incongruenza nella dichiarazione della loro inammissibilità da parte della Commissione.

Signor Presidente, illustro gli emendamenti 2.111 e 2.186, che si riferiscono alla Pedemontana lombarda e alle connesse tangenziali di Como e Varese. Com'è noto, questa è un'opera attesa da decenni dalle province lombarde, presente nell'allegato infrastrutture di Milano Expo

lo dico perché abbiamo votato in Commissione un ordine del giorno unitario (sostenuto da maggioranza e minoranza) che dà priorità alle opere cantierabili nel 2009

sul 2.350, che risponde all'esigenza - manifestatasi, purtroppo, in maniera tragica - di interventi per le spese finalizzate alla messa in sicurezza degli istituti scolastici. questione propone che ciò si possa fare direttamente da parte degli enti locali, con una deroga alla contabilizzazione di quelle spese nel Patto di stabilità. Gli enti locali - e lo dico per esperienza diretta hanno numerose risorse per avanzi di amministrazione che non possono spendere per nessun motivo. Ora, esentarli dal computo del Patto di stabilità per le spese finalizzate alla messa in sicurezza degli istituti scolastici credo credo possa risolvere anche il problema di stanziamenti notevoli, che diversamente lo Stato dovrebbe andare ad affrontare in maniera diretta. Qualcuno potrà eccepire che i precedenti stanziamenti statali non sono stati tutti utilizzati ma chi ha esperienza di questa vicenda sa bene che essi non sono stati utilizzati per il filtro - a mio giudizio, assolutamente anomalo e non corrispondente allo spirito del Titolo V della Costituzione - che le Regioni hanno imposto nell'utilizzazione di queste cifre stanziate dallo Stato e destinate agli enti locali. Buona prassi vorrebbe che questi fondi andassero direttamente agli enti locali, perché è dimostrato che il filtro regionale crea una vischiosità nell'utilizzo di queste somme, rendendole poi in parte anche inefficaci. L'emendamento 2.399 risponde ad un'esigenza precisa, relativa ai Comuni che stanno provvedendo - faticosamente, lo sappiamo - alla ricostruzione dopo il terremoto del Belice, e non comporta alcuna spesa. È infatti impropria l'aggiunta della copertura, poiché in una riunione con il Ministro per la semplificazione che occorreva ripristinare alcuni numeri dell'allegato A del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, che ha previsto l'abolizione di una serie di norme, tra le quali quelle indispensabili per l'operatività dei Comuni, su fondi già assegnati.

Spero che il rappresentante del Governo abbia voluto al riguardo compulsare il Ministro della semplificazione che in più di un incontro ha detto che assolutamente questa norma andava ripristinata. Infine, gli emendamenti 2.6120 e 2.6121, signor Presidente, rispondono all'osservazione all'unanimità fatta sul testo della legge finanziaria dalla Commissione ambiente che ho l'onore di presiedere: in quella osservazione, infatti, la Commissione ha ritenuto di dovere rilevare che, mentre i fondi destinati alla tutela ambientale, di cui all'articolo 1, comma 432, della legge n. 266 sono stati decurtati di quasi il 50 per cento e quindi di oltre 250 milioni (su questo, se le esigenze di bilancio lo impongono, pazienza, *nulla quaestio*), in corrispondenza è stato incrementato il Fondo ad eguale destinazione per gli interventi sull'ambiente presso il Ministero dell'economia e finanze. Alla Commissione è parsa assolutamente strana la prassi

vorrà considerare l'opportunità dell'osservazione fatta dalla Commissione ambiente e dare anche a questa osservazione un suo riscontro. Diversamente, signor Presidente, le Commissioni producono condizioni, osservazioni e suggerimenti ai disegni di legge *in itinere*, ma poi, vedendoli disattesi, potrebbero anche decidere un domani di non produrre più in quanto ritenuti assolutamente ultronei. *(Applausi del

sul cui territorio sono ubicati impianti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali e GPL, nonché impianti per la produzione di energia elettrica, possano avere una compartecipazione alle accise che tali impianti versano allo Stato nella misura determinata nell'1 per cento, a seconda della popolazione che risiede in quel territorio. Naturalmente, tutto questo con finalità di tipo ambientale perché ovviamente questi Comuni, sedi di raffinerie o di impianti di questo tipo, subiscono un'alterazione ambientale e i cittadini pagano anche le conseguenze per avere l'ubicazione di questi impianti. Secondo l'emendamento, queste somme sono quindi prioritariamente destinate alla gestione del territorio, anche in relazione alla presenza di queste attività produttive, ed in particolare ad opere di viabilità, di controllo dell'urbanizzazione, di realizzazione di infrastrutture e sopratutto di tutela ambientale. Credo che, in un'ottica in cui guardiamo ai Comuni con una sensibilità nuova, visto e considerato che tanti tagli sono fatti, almeno per questi Comuni debba essere previsto un aiuto da parte dello Stato, favorendo la compartecipazione alle accise. Di analogo tenore, signor Presidente, anche se un po' diverso, è l'emendamento 2.153.

naturalmente non è stata mai applicata, perché non sono mai stati emanati, d'intesa con la Conferenza unificata, i decreti attuativi per poterla rendere operativa. È stata resa operativa soltanto per la Sicilia; quindi, tutto ciò comporta anche una disparità di trattamento assolutamente inaccettabile, perché gli impianti di raffinazione e di stoccaggio di oli minerali e di gas sono presenti in diverse parti d'Italia. Per tale ragione chiediamo venga data attuazione a questa norma, che è rimasta ancora oggi lettera morta.

che quindi vengono presi in carico dalle strutture di assistenza comunale, non riescono più a far fronte alle spese e agli oneri che comportano l'assistenza e l'integrazione di questi ragazzi, anche al fine di dar loro una tutela sotto il profilo della salute fisica, nonché la consapevolezza di doversi integrare nella comunità e frequentare la scuola. Per questo motivo a tali Comuni si vorrebbe destinare una quota pari a 10.000 euro per ciascun minore, da utilizzare per l'attuazione delle misure di assistenza, accoglienza, integrazione ed eventuale ricongiungimento con i rispettivi genitori. Credo che nell'ottica delle politiche che il Governo ha più volte sottolineato e propagandato tale emendamento possa e debba essere accolto. Infine, signora Presidente (gradirei che la signora Presidente mi ascoltasse,

*(PD)*. Signora Presidente, do per illustrato l'emendamento 2.149, avente per oggetto l'accisa sul gas metano per le Province di Aosta, Belluno, Bolzano, Sondrio e Trento, nelle quali oltre il 70 per cento dei Comuni ricade nella zona climatica F. Do altresì per illustrato l'emendamento 2.0.10, avente ad oggetto il contributo dovuto al Servizio sanitario nazionale per le prestazioni erogate ai cittadini coinvolti in incidenti di veicoli a motore o di natanti. l'emendamento 2.401. L'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 279 del 1974, recante norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di minime proprietà colturali, caccia e pesca, agricoltura e foreste, prevede, ai fini della valorizzazione delle zone montane, che le Province autonome possano costituire tra i Comuni appartenenti ad uno stesso comprensorio, le comunità montane previste dalla legge 3 dicembre 1971, La Provincia autonoma di Trento ha recentemente riorganizzato il sistema delle istituzioni provinciali e locali con legge provinciale n. 3 del 2006, recante norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino. Nell'ambito di tale disciplina, è prevista, tra l'altro, l'istituzione di enti pubblici, denominati comunità, costituiti dai Comuni appartenenti al medesimo territorio per l'esercizio di funzioni, compiti, attività e servizi, nonché in forma associata obbligatoria delle funzioni amministrative trasferite ai Comuni, secondo quanto disposto dalla medesima legge provinciale. La proposta di emendamento 2.401 è diretta a chiarire che anche le comunità istituite ai sensi della predetta legge provinciale rientrano tra i soggetti ai quali non si applica l'imposta in estensione delle previsioni di enti pubblici elencati nel primo comma dell'articolo 74

nel modo dovuto in questa fase la necessità di sostenere il risparmio energetico per le imprese che operano in questo settore, così come per i cittadini che vogliono ottenere un risparmio energetico. Potrebbe essere un'utile correzione di rotta,

L'emendamento 2.513 richiama invece la necessità di strutturare in termini manageriali le piccole e medie imprese del Mezzogiorno del Paese.

Ricordo in sintesi le questioni: la questione energetica e il tema delle energie rinnovabili, lasciando sullo sfondo la questione dei cambiamenti climatici, e la questione del trasporto pubblico, con il connesso tema del pendolarismo e dei contratti di servizio

produrre almeno il 20 per cento dell'energia con fonti rinnovabili, aumentare del 20 per cento l'efficienza energetica rispetto alle proiezioni del 2020, ridurre del 20 per cento le emissioni di gas serra rispetto ai livelli del 1990. Dove vuole fermarsi l'Italia?

spenderci sulle energie alternative e sulla limitazione virtuosa dei consumi energetici. Qualcosa in tal senso si poteva fare. Immaginare un sistema di incentivi, peraltro spesso già previsti in passato, sia per la produzione di energia elettrica da fonte alternativa, sia per sostenere consumi buoni delle famiglie con ecoincentivi per gli acquisti di elettrodomestici a consumi più contenuti sarebbe saggio. Perché allora non pensarci? In tal senso si collocano, ad esempio, alcuni emendamenti come il 2.167 e il 2.168. La seconda questione che vorrei ricordare riguarda la stipula dei contratti di servizio dello Stato e delle Regioni a Statuto ordinario con Trenitalia Spa per la fornitura dei servizi ferroviari regionali. Si tratta dell'emendamento 2.257. Non ho bisogno di ricordare in questa sede il fenomeno del pendolarismo: 14 milioni di persone al giorno che si spostano in Italia, di cui 2 milioni con il trasporto in treno. Non serve forse neanche ricordare le disagiate e quasi inumane condizioni dei viaggiatori pendolari, costretti a viaggiare su materiale vecchio, sporco, in pessime condizioni, con ritardi, al freddo o al caldo eccessivo. Tali viaggiatori spesso sono anche costretti a fare i conti con la soppressione dei treni. Inutile ricordare ancora come il trasporto di questo tipo, ossia su treno, evita un ulteriore aggravarsi del traffico veicolare su strade e autostrade; traffico che, soprattutto in prossimità dei centri urbani, è spesso insostenibile oltre

ha provocato un esodo silenzioso, ma continuo, verso i territori delle Province e verso le periferie. Da lì la gente deve tornare a rifluire sulla città per il lavoro

corollario necessario sui temi della mobilità alternativa, a cui era dedicato anche l'emendamento 2.112 appena citato, finalizzato alla valorizzazione e allo sviluppo della mobilità ciclopedonale.

Avremmo desiderato che non si perdesse un'ulteriore occasione in tal senso, soprattutto quando altri Paesi europei, come la Francia ad esempio, sembrano muoversi più speditamente di noi. Per questo motivo ci auguriamo che i nostri emendamenti vengano votati, perché non vorremmo che il Paese perdesse su questi temi l'ennesima occasione.

per quanto riguarda il Veneto, nel 2009 sono state azzerate in maniera drastica le risorse destinate alle infrastrutture. Varrebbe la pena ricordare anche solo le opere di integrazione del Passante, le opere del porto di Chioggia, il riequilibrio idrogeologico della laguna, i fondi dell'ANAS

Va ricordato anche che il sistema ferroviario metropolitano regionale prevede una serie di treni regionali ad elevata frequenza e ad orario cadenzato e un sistema di mobilità avanzato che è imperniato su tre poli principali, quali Venezia, Padova e Treviso, e su una serie di poli secondari. Quindi, il completamento di questo progetto potrebbe garantire livelli di integrazione territoriale e di prestazioni di trasporto adeguati al tessuto industriale e alla mobilità sociale di un'area strategica del territorio nazionale che concorre - lo ricordo - alla formazione del prodotto interno lordo del Paese con una quota del 9,4 per cento e che è seconda solo alla Lombardia. milioni di euro che erano stati stanziati dalla legge finanziaria per il 2008 erano parte essenziale di quei 140 milioni di euro necessari al completamento delle tratte del sistema metropolitano ancora non finanziate:

del Fondo per gli ex esposti ad amianto, la bonifica di siti e immobili inquinati da amianto e la sorveglianza sanitaria di coloro che hanno risentito degli effetti negativi dell'esposizione all'amianto Ricordo, in particolare per il Ministero del lavoro, che già con la passata legge finanziaria per il 2008 era stato istituito un Fondo per gli ex esposti all'amianto e per le vittime dell'amianto e che questo fondo è ancora bloccato a seguito dell'omissione

nel computo dei risultati del patto di stabilità interno delle Regioni e delle Province autonome anche quelle spese in conto capitale per interventi cofinanziati dall'Unione europea e non per la parte di competenza regionale. Questa modifica consentirebbe a molte Regioni - non soltanto a quelle del Mezzogiorno, ma in modo particolare a quelle - la chiusura dei programmi comunitari e consentirebbe a tanta parte del nostro territorio di vedere garantito il finanziamento dei progetti d'investimento e di sviluppo.

che non ci sono, dall'altra, con questa norma - se non corretta - vanifica la possibilità di utilizzare gli investimenti e i finanziamenti già disponibili, che servono allo sviluppo di tanta parte del nostro territorio.

il meccanismo del credito d'imposta, ovvero di far ricorso all'automatismo dell'incentivazione alle imprese che realizzano investimenti. Con lo stesso emendamento provvediamo ad aumentare la disponibilità di risorse, che è stata fortemente decurtata. Come i colleghi sanno, ad uno strumento unanimemente apprezzato negli anni passati dall'intero sistema imprenditoriale e dalle sue stesse rappresentanze associative per aver unito la certezza delle risorse a seguito della realizzazione degli investimenti all'efficacia delle procedure, con una snellezza all'insegna dell'automatismo. In tal modo si sono superate - a onor di cronaca è giusto ribadirlo in questa sede - le pastoie burocratiche, spesso sfociate in forme di inquinamento e di distorsione nell'utilizzazione delle risorse pubbliche, cui hanno dato vita altri strumenti di incentivazione come, ad esempio, la legge n. Insomma, si tratta di uno strumento che negli anni trascorsi ha dato certezza per le strategie di investimento delle imprese, in particolare nel Mezzogiorno d'Italia. Oggi questa certezza è venuta meno, a seguito dell'introduzione di una serie di procedure che hanno messo in discussione il meccanismo dell'automatismo, procedendo anche ad una forte decurtazione delle risorse disponibili. L'emendamento affievolisce il ripristino *tout court* dello strumento com'era prima dell'intervento legislativo cui il Governo ha dato seguito con il decreto-legge n. n. 97. Quella scelta è stata spesso motivata da parte del Governo, e del ministro Tremonti in particolare, con la necessità di effettuare un monitoraggio nell'uso delle risorse pubbliche. Se questa è la motivazione, possiamo convenire e proponiamo con questo emendamento che a tale monitoraggio si possa ricorrere in corso d'opera, attraverso una verifica nel prossimo triennio che culmini in un momento d'incontro tra i Ministeri interessati, in particolare il Ministero dello sviluppo economico, e le forze sociali, a cominciare da quelle imprenditoriali e sindacali,

Auspichiamo che su questa necessità, che molte organizzazioni imprenditoriali (tutte vorrei dire) e l'intero sistema delle imprese hanno manifestato nelle scorse settimane, levando una voce di vibrata protesta protesta contro l'intervento che vuol mettere in discussione e sostanzialmente annullare l'efficacia dello strumento del credito d'imposta, vi possa essere un'attenzione da parte del Governo e della maggioranza. Faccio ovviamente appello innanzitutto alla coerenza

unanimemente riconosciuta dello strumento in oggetto. Mi auguro dunque che si possa tornare all'apprezzato strumento del credito d'imposta, così com'è stato utilizzato, nei mesi e negli anni passati, dall'intero sistema imprenditoriale del Paese e in particolare delle aree svantaggiate.

Presidente, la criminalità organizzata e le mafie utilizzano il racket e l'usura come una sorta di bancomat per le loro attività criminali.

2.282 chiediamo che la discussione sul trattamento economico accessorio per i dipendenti della pubblica amministrazione avvenga previa intesa con le organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, perché

che aveva regolamentato in modo penalizzante il trattamento economico accessorio per la pubblica amministrazione. Si chiede perciò di tornare alla precedente disciplina. Voglio solo ricordare, ad esempio, che all'articolo 67,

onorevoli senatori, intervengo per illustrare l'emendamento 2.254 relativo alla specificità dei compiti e dei doveri delle Forze armate e delle Forze di polizia. Il Parlamento ha già riconosciuto questa specificità e tale riconoscimento, mi sembra di poter dire, è generalmente e fortemente condiviso dagli onorevoli senatori. Ne sono testimonianza le espressioni di apprezzamento che i rappresentanti sia della maggioranza che dell'opposizione hanno più volte indirizzato agli uomini e alle donne in uniforme per la loro professionalità e il loro impegno. Ne sono testimonianza, soprattutto, il sincero cordoglio e la forte vicinanza alle famiglie che la Presidenza del Senato e tutti i Gruppi parlamentari hanno manifestato verso le Forze armate e di polizia nei casi, purtroppo frequenti, in cui l'assolvimento dei loro compiti e il rispetto dei loro doveri hanno comportato il sacrificio della vita da parte di taluni appartenenti a quelle forze. signori senatori, l'emendamento 2.254 cerca di interpretare proprio questo sentire, che è comune in quest'Aula ma è comune soprattutto nel Paese, vuole evidenziare l'attenzione nei confronti di una categoria che svolge una funzione insostituibile per la tutela delle istituzioni, la salvaguardia e la sicurezza in Italia e all'estero. si rivolge ad un'entità numerosa, ai 500.000 operatori del comparto difesa e sicurezza e alle loro famiglie.

contenuta, ma più presentabile di quella - lasciatemelo dire - piuttosto imbarazzante di tre euro al mese mese attualmente prevista negli stanziamenti forniti dal Governo. Mi auguro, quindi, che tutti i colleghi senatori vogliano sostenere l'approvazione di questo emendamento e mi auguro che il Governo voglia cogliere questa opportunità opportunità dando, sia gli uni che l'altro, un segno tangibile della stima e dell'apprezzamento che nutrono verso le Forze armate e le Forze di polizia.

la nostra Capogruppo, senatrice Finocchiaro, elencando nella sua dichiarazione di voto le ragioni che ci vedevano fortemente contrari, ne ha sottolineate soprattutto due:

la stessa sollecitudine che abbiamo visto nei confronti dell'appello dei vescovi vorrà trovare un altrettanto sollecito riscontro anche negli emendamenti che abbiamo depositato, cogliendo il grido di dolore della scuola pubblica.

Presidente, intervengo sempre in tema di scuole e caserme per ricordare l'assoluta necessità di ripristinare la dotazione di un fondo soppresso dal decreto-legge

centinaia di plessi scolastici sparsi sul territorio nazionale e degli appalti di pulizia e ristorazione in decine di caserme sul territorio nazionale. Tali appalti vengono resi grazie all'intervento di alcune decine di imprese raggruppate in consorzi, molte delle quali, in assenza del ripristino dei fondi, si troveranno del tutto prive di attività e quindi dovranno chiudere; corrispondono complessivamente all'occupazione di 15.000 lavoratori per le scuole e di 8.000 lavoratori per le caserme. Per tutti costoro sono già state avviate dalle imprese titolari degli appalti le procedure di mobilità. Il decreto-legge n. 185 all'esame della Camera dei deputati stanzia per le sole scuole 110 milioni di euro, che sono l'equivalente di circa un quarto delle risorse necessarie a garantire la prosecuzione

Noi abbiamo proposto delle misure diverse e realizzabili. Ci sono due emendamenti che ho presentato a tale proposito (il 2.426 e il 2.428) che ci aiutano ad incrementare

con uno spostamento della base produttiva del Paese verso aree sottoutilizzate e con la possibilità, in questa fase di crisi, di dare incentivi finalmente qualificati e finalmente in grado di produrre dei veri risultati.

il tema delle accise sui prodotti petroliferi. Ebbene, la proposta che avanziamo è quella di rendere finalmente

prodotti petroliferi in termini di trasformazione e di raffinazione e per quanto riguarda la benzina senza piombo ed il gasolio per autotrazione,

sono poi una serie di emendamenti, uno in particolare sulla viabilità minore, che è stata scippata scippata dal Governo di centrodestra all'utilizzo per una infrastrutturazione in grado di produrre utilità nel sistema viario e anche una ricaduta positiva in termini economici.

con delle risorse che spesso non sono utilizzate e che spesso sono ancora nelle mani delle cosche mafiose.

Con questo comma si impone la riduzione di 10 milioni di euro, da 55 a 45, dell'importo complessivo dei contributi che possono essere concessi in favore dei piccoli Comuni con popolazione residente ultrasessantacinquenne particolarmente elevata, per stornarli in favore dei piccoli Comuni con popolazione residente al di sotto dei cinque anni molto elevata. Oltre allo spostamento di risorse, di fatto con tale opzione si afferma un metodo di scelta inaccettabile sul piano della civiltà, quello dello scontro fra generazioni. È un metodo che ricorda certe abitudini tribali che imponevano la morte degli anziani nei momenti di carestia. Questo comma, con le scelte e soprattutto con il metodo che sottintende, non tiene conto degli andamenti demografici, delle loro conseguenze e della necessità di di sostenere diversificate politiche per l'invecchiamento attivo: non solo per ragioni di inclusione sociale e di civiltà ma per la necessità di effettuare adeguati investimenti per evitare, nel prossimo futuro, conseguenze devastanti su altri rilevantissimi equilibri economici quali l'assistenza, le pensioni e la sanità. Gli andamenti demografici ci richiedono di sostenere tutte quelle iniziative utili a sostenere l'autonomia dell'anziano e a ridurre i tempi di cura. Tali necessità, proprio a partire dall'analisi sull'invecchiamento della popolazione, sono ampiamente rilevate dalla Comunità europea che indica, nel sostegno alle politiche di *active aging*, uno dei futuri perni per uno sviluppo sociale ed economico civile e sostenibile. Scelte di questo tipo, ancorché non impossibili, andrebbero tuttavia collocate in ambiti diversi e, soprattutto, dovrebbero essere sostenute da valutazioni molto più generali e approfondite. valutazioni, riferendosi allo specifico provvedimento, rientra anche l'aver ben presente cosa si voglia fare per la sopravvivenza e la qualità della vita dei piccoli insediamenti urbani. Tali ragionamenti, comunque, in nessun caso dovrebbero essere svolti basandosi sul principio della contrapposizione generazionale. Per questo motivo, ritengo che questo comma 40 non abbia alcuna giustificazione: né demografica, né sociale né, tanto meno, economica.

Signora Presidente, illustrerò una serie di emendamenti relativi al Patto di stabilità per gli enti locali. Questi emendamenti si collocano all'interno della manovra espansiva, proposta dal Partito Democratico, che i caratteri efficacemente illustrati dal senatore Morando. È una manovra volta al sostegno del reddito delle famiglie (quindi alla domanda interna) e al sostegno degli investimenti, partendo da quelli pubblici. Io mi riferisco in particolare agli investimenti degli enti locali. Gli emendamenti riguardano i Comuni virtuosi, quelli che hanno rispettato il Patto di stabilità; stabilità; le risorse che provengono a questi Comuni da utili di partecipazione azionaria (ad esempio, di società di gestione di servizi pubblici locali); le risorse proprie derivanti da gestioni dirette di servizi a rilievo economico; ancora, le risorse provenienti dall'Unione europea che necessitano di cofinanziamenti da parte degli enti locali; le risorse esistenti, disponibili, non provenienti da prelievi fiscali ma non spendibili a causa del vincolo del vincolo del Patto di stabilità, bloccate e quindi incapaci di generare investimenti, produzione, occupazione e domanda interna. Noi indirizziamo questo allentamento dei vincoli a destinazioni specifiche, a investimenti e, in particolare, la mia proposta è per realizzare investimenti in infrastrutture e investimenti per la sicurezza delle scuole e per l'edilizia scolastica mirata appunto alla sicurezza. Un ulteriore emendamento che voglio illustrare è teso a rendere più efficace e più efficiente la gestione dei servizi da parte degli enti locali: emendativa 2.339, che prevede un incremento del fondo a sostegno della gestione associata dei servizi e delle funzioni comunali, naturalmente in riferimento a quei piccoli Comuni per i quali sosteniamo fortemente le unioni comunali, perché questa gestione dei servizi sia maggiormente efficace ed efficiente.

alle spese relative alla messa in sicurezza degli edifici scolastici. Il Governo Berlusconi per il 2009 ha tagliato 22,8 milioni di euro sugli investimenti in sicurezza scolastica e l'emendamento vuole intervenire su quest'assurda situazione. signor Presidente, che, soltanto nel pomeriggio di oggi, una scuola elementare di Roccaraso in Abruzzo è stata velocemente evacuata perché un ingegnere scrupoloso e attento,

escludere dai vincoli del Patto di stabilità interno le spese sostenute dalle Regioni e dagli enti locali per le opere di intervento di messa in sicurezza e di adeguamento degli edifici. Tenga conto, signor Presidente, che, di fronte a tale proposta, come ad altre che sono state illustrate dai miei colleghi

s'intende intervenire su una questione già sottoposta all'attenzione di quest'Aula, quando, con la finanziaria del 2008, venne approvato un investimento di 168 milioni di euro in infrastrutture, per la linea ferroviaria Roma-Pescara, una delle più vetuste che esistano nel nostro territorio nazionale, utilizzando il FAS: finalmente, ciò per cui occorrono i fondi che sono stati saccheggiati dal Governo Berlusconi. È molto strano, ma anche su questi emendamenti il Governo, insieme al relatore, ha espresso parere contrario. Eppure, signor Presidente, il nostro presidente del Consiglio Silvio Berlusconi si è recato in Abruzzo negli ultimi due fine settimana e ha parlato di 19 miliardi di euro da investire in infrastrutture; ma - guarda caso - quando abbiamo proposto emendamenti di valore molto, molto inferiore su tre cifre diverse, proprio affinché il Governo e il relatore potessero scegliere quale carta utilizzare e giocare), hanno detto di no a tutto. andava da un emendamento radicale di 400 milioni di euro per un anno, passando per uno di 200 milioni di euro per tre anni, ad un altro di 56 per tre anni, com'era nella finanziaria. Eppure, signor Presidente, qualche emendamento di questi era stato sottoscritto da parlamentari della destra, ancorché non abruzzesi (visto che, tranne il senatore Pastore, sempre presente in Aula, altri della destra non sono stati mai presenti né in Commissione bilancio né tanto meno in quest'Aula).

negativo da parte di quest'Aula - sui fenomeni di emergenza dei quali ci si occupa fra i mesi di aprile e maggio, sapendo che scoppieranno a luglio ed agosto (ma, quando si ha la possibilità di occuparsene per tempo, ci si rifiuta di intervenire). in queste aree, come ad esempio quella del Fucino in Abruzzo o altre viciniore, c'è un bisogno essenziale, visto che da trent'anni non si realizzano opere di alcun tipo per migliorare il piano idrico. In ultimo, signor Presidente, illustro l'ordine del giorno G3.138 che riguarda il 5 per mille. Non abbiamo visto nella finanziaria né in altri documenti che riguardino la reintroduzione di quanto previsto nella legge finanziaria 2008, già previsto nella legge finanziaria 2007, cioè una disciplina finanziata da questo Governo per l'anno in corso, nell'ambito della sua legge finanziaria, volta a prevedere la possibilità di destinare il 5 per mille dell'IRPEF a finalità di sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale. È evidente che questo argomento non interessa

per la messa in sicurezza degli edifici scolastici. Quando successe il grave fatto di Torino, il Ministro dell'istruzione assicurò assicurò che il Governo sarebbe intervenuto efficacemente in materia; anzi, accusò l'opposizione di speculare su questa tragedia solo per il fatto che l'opposizione esponeva i dati di fatto, cioè i pesanti tagli di bilancio che sul piano degli investimenti per l'edilizia scolastica venivano praticati. C'è il momento delle parole e vi è sempre il momento dei fatti: quello del bilancio è sempre un momento dei fatti.

nel 2009 del 37 per cento, signor Sottosegretario, e addirittura nel 2010 rispetto al 2009 dell'82 Con quale faccia il Ministro si presenta di fronte al mondo della scuola sostenendo che farà tutto il possibile per la buona manutenzione degli edifici scolastici con tagli di questa dimensione? Noi proponiamo intanto una strada semplice. Gli enti locali hanno a disposizione delle risorse. Come ha riconosciuto anche il sottosegretario Vegas, sarebbero risorse che possono trovare rapidamente impiego nel ciclo economico. Non si capisce perché non si debba accogliere questo ed altri emendamenti che consentono agli enti locali di avviare questo ciclo di investimenti. Cosa costerebbe questa esclusione? Costa un quinto di quanto il Governo ha riservato come regalo al Comune di Catania; un quinto del costo della mancia al Comune di Catania per consentire a tutti i Comuni italiani di di intervenire in questa materia. Mi domando se vi è una qualsiasi ragione per dire di no ad un emendamento di evidente buonsenso.

gli obiettivi politici di cui alla tabella C? Non ho mai visto un taglio di 400 milioni e ne rimangono meno di quelli tagliati: Chiedo perché non si cancella tutto quanto il capitolo. Se c'è una critica da fare alla cooperazione allo sviluppo si abbia il coraggio di cancellare quella legge, ma, se si vuole mantenere una legge in quelle condizioni, la mia domanda è: chi decide chi decide gli obiettivi politici, il Ministero degli affari esteri o il Ministero dell'economia? Credo che le salmerie dovrebbero essere quelle del Ministero dell'economia. Liberiamoci, votando questo emendamento, dall'idea che la politica debba seguire l'economia.

della Dichiarazione universale dei diritti umani e tale emendamento riguarda l'adeguamento del fondo per le vittime della tratta degli esseri umani. Se non si coglie questa occasione, due sono le conseguenze che si debbono trarre: in primo luogo, che noi vogliamo continuare a violare i diritti umani (e ci dobbiamo occupare dei diritti umani violati in Italia oltre che all'estero); in secondo luogo, che non vogliamo seriamente portare avanti un programma in materia di sicurezza. Sostenere infatti le vittime del traffico di esseri umani attraverso programmi di assistenza significa sostenere i processi contro i trafficanti di esseri umani, che sono di competenza delle procure distrettuali, che, difatti, da questi interventi in materia di tratta, che il Dipartimento per le pari opportunità ha cofinanziato (fino a 533 progetti per 54.559 vittime), hanno tratto grandissimo vantaggio per i processi. Quindi, se tale emendamento non passerà, vi è un difetto di coerenza del Governo e della maggioranza.

accessibile) possa esserci una convergenza, non soltanto dell'opposizione ma anche della maggioranza.

all'abolizione dell'ICI. Chiediamo il ripristino di questi fondi, che in parte dovrebbero essere destinati anche al finanziamento delle accademie non statali: Perugia, Genova, Bergamo, Brescia e Ravenna, che attualmente versano in una situazione di grave crisi economica.

Sottolineando, quindi, l'importanza dell'alta formazione artistica e musicale, quale veicolo della tradizione e della cultura italiana nel mondo, e nell'attesa della statalizzazione delle accademie attualmente non statali, chiediamo che si dia seguito all'impegno preso con quell'ordine del giorno stanziando adeguate risorse per sostenere questi enti. Signor Presidente, rappresentanti del Governo, onorevoli senatrici e senatori, l'emendamento 2.545 mira ad introdurre criteri moderni, riconosciuti a livello internazionale, per l'assegnazione dei fondi pubblici per la ricerca. Attualmente la situazione italiana si può riassumere in tre concetti: fondi assolutamente insufficienti, controllati da pochi; assenza di trasparenza; meritocrazia. La meritocrazia è un sistema di governo dell'azione collettiva basato sull'abilità dimostrabile e sul talento, piuttosto che sulle relazioni familiari e clientelari, sul nepotismo o su privilegi di posizione sociale. La situazione italiana è l'opposto, fatto che ci impoverisce e spinge i nostri cervelli migliori a emigrare all'estero. Non si può più tollerare quest'anomalia e non ci si può comportare come se fosse un destino ineluttabile. E, infatti, non lo è. Ne abbiamo avuto la prova recentemente, con un concorso pulito che ha portato all'assegnazione di 16 milioni di euro a 26 giovani ricercatori con meno di 40 anni, selezionati con il sistema della *peer review* da una commissione di dieci membri anch'essi con meno di 40 anni. Ognuno dei vincitori ha adesso a disposizione 600.000 euro per tre anni e potrà dimostrare quanto vale. Sapete chi si è aggiudicato il primo posto tra i 1.720 progetti presentati a questo concorso? Una ragazza di Chieti, di trent'anni, con un progetto di ricerca sulle malattie neurodegenerative, una ragazza che era stata recentemente scartata nella sua università quando aveva partecipato ad un concorso per un posto da ricercatrice. È l'ennesima prova che il sistema attuale non è in grado di selezionare e promuovere chi dimostra creatività e impegno. Le difficoltà dell'Italia nel destinare fondi adeguati alla ricerca e nell'adottare un sistema di valutazione trasparente sono sotto gli occhi di tutti; riviste scientifiche internazionali come "*Nature*" e "*Science*" pubblicano in questi giorni editoriali critici e preoccupati. Ma se non si è pensato ad aumentare la quota degli investimenti, pensiamo almeno a distribuire i pochi fondi in maniera intelligente. Introdurre la *peer review*, il giudizio tra pari, e abbandonare l'assegnazione discrezionale dei fondi pubblici è un passo necessario. È un metodo sperimentato e adottato dalla comunità scientifica internazionale, auspicato dai nostri ricercatori e anche dalla realtà industriale italiana, come ha ribadito di recente anche Sergio Dompé, presidente Anche il sottosegretario Fazio ha sostenuto in varie occasioni la necessità dì introdurre regole rigide, meritocrazia, trasparenza. Tutti princìpi assolutamente giusti, ma che nella pratica non si vedono ancora applicati. prese invece decisioni in controtendenza con le scelte delle principali democrazie occidentali. La Svezia, partendo da finanziamenti pari al 3,9 per cento del PIL, ha varato un piano massiccio di investimenti in innovazione e ricerca contro la crisi economica; lo stesso ha fatto la Francia, che ha raddoppiato gli investimenti. Tutte le principali Nazioni dell'Europa occidentale marciano speditamente verso il 3 per cento del PIL investito in ricerca. Il Governo italiano ha scelto invece la strada inversa: ridurre i già magri fondi per la ricerca e passare dall'1,1 per cento Di fronte a questa situazione è nostro dovere introdurre il criterio del merito: occorre garantire per legge che nessun soldo proveniente dalle tasse dei cittadini sia mai più erogato senza *peer review* e che nessuna finanziaria possa assegnare milioni di euro a istituzioni di ricerca o ricercatori senza prevedere alcuna competizione, come succede ora. Mi rivolgo ai senatori della maggioranza con cui abbiamo lavorato per andare in questa direzione. Mi rivolgo ai senatori Tomassini, Cursi e Pisanu: in passato abbiamo apprezzato la vostra serietà e determinazione e sono certo che anche voi ricorderete gli sforzi che abbiamo compiuto assieme nella direzione di premiare i migliori. Vi chiedo di sostenere assieme l'opportunità di dare a questo Paese delle regole moderne, indispensabili per far progredire gli scienziati più capaci e le idee più promettenti. Dimostriamo con il voto di tutti che questo Senato, nel gestire i fondi pubblici, non vuole il modello dell'università di Messina, ma vuole invece scardinare il sistema di potere dei baroni e degli amici degli amici. Votiamo assieme un emendamento che - lo voglio ricordare -, non implicando maggiori spese a carico dello Stato, permetterà tuttavia di modificare radicalmente un sistema corrotto che ha bisogno di correttivi urgenti. Restituiamo con il nostro voto la speranza a chi crede nella meritocrazia.

Signora Presidente, l'emendamento 2.503 si propone di disporre l'esenzione delle accise sulle benzine, sul gasolio e sul gas

il Senato ha già espresso un orientamento attraverso il voto su un ordine del giorno, approvato anche dalla maggioranza, con il quale il Governo confermava l'annuncio già formulato in circostanze precedenti circa l'adozione di tale provvedimento. Ci pare sia giunto il momento di operare in maniera coerente con gli annunci effettuati. Con l'emendamento 2.549 torniamo sul tema dell'edilizia scolastica. Già è stato detto molto in relazione all'esigenza di attivare le procedure più efficaci perché l'edilizia scolastica possa presentare quelle necessarie e indispensabili garanzie di stabilità e di sicurezza, anche per l'impatto che ciò determina sulla tranquillità e sui fattori di civiltà che noi dovremmo rivendicare a partire dai luoghi di formazione dei cittadini del domani, di trasmissione della conoscenza e del sapere. In aggiunta a tutto ciò, proponiamo di utilizzare strumenti e conoscenze già oggi disponibili e nella disponibilità del Dipartimento della protezione civile,

un patrimonio di regole, di procedure, di specifiche funzionali ed operative, validate non solo dalla comunità scientifica, ma fatte proprie dal Dipartimento della protezione civile, perché tutte le attività e le risorse spese in questo settore possano essere qualificate dal punto di vista dell'efficacia e dell'efficienza. La nostra proposta, dunque, è di fissare un percorso operativo

in una situazione di scarsezza di risorse finanziarie; non solo, ma anche per determinare quella virtuosità degli interventi che possono restituire anche benefici in termini di finanza pubblica. agendo per la messa in sicurezza impiantistica e per l'efficienza energetica, si attivano quelle operazioni in grado di restituire benefici sulle partite correnti e, quindi, sui costi operativi delle pubbliche amministrazioni.

una norma con la quale si consentiva ai soggetti colpiti dalle alluvioni del novembre del 1994 di definire in via automatica la propria posizione tributaria relativamente agli anni 1995, 1996 e 1997,

Il problema è che soprattutto l'INPS si è sempre rifiutato di applicare la legge. Nonostante il difensore civico del Piemonte e il garante del contribuente avessero dato un'interpretazione conforme alla volontà reale del Parlamento, l'orientamento dell'INPS è stato sempre quello di non accogliere le domande. Fortunatamente, è stato poi approvato un emendamento, presentato dal Gruppo della Lega Nord Padania

inequivocabile della norma. Faccio presente che l'ultima decisione di portare in causa un contribuente era firmato Mastrapasqua che è il neoeletto presidente dell'INPS. Direi che siamo veramente al ridicolo.

Con tutta una seria di iniziative ed alcune proroghe, nelle varie finanziarie riuscimmo ad evitarlo; dopo di che, con altre iniziative, facemmo in modo che

che questo problema debba essere risolto con un disegno di legge, perché riguarda anche coloro che sono in stato di quiescenza e che continuano a pagare trattenute pesanti per il fisco: io stesso

ordine del giorno, che riguarda la formazione professionale iniziale che era stata potenziata dal Governo Berlusconi nella XIV legislatura, autorizzando i percorsi sperimentali di durata triennale, ed è stata rimodulata dallo scorso Governo Prodi, che aveva introdotto l'obbligo di istruzione e di prosecuzione dei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale fino alla messa a regime dell'obbligo

perché permette di assolvere l'obbligo di istruzione non solo nel sistema scolastico, ma anche in quello formativo, collocando la scelta della formazione professionale al termine della scuola media e non come ripiego al fallimento scolastico. Non a caso dal 2003 ad oggi il numero degli allievi che ha optato per questa scelta è progressivamente aumentato, fino a raggiungere la cifra di 110.000 circa. Togliere alle nostre ragazze e ai nostri ragazzi questa opportunità significa privarsi anche della funzione di contrasto alla dispersione scolastica. Per questo motivo chiediamo che il Governo si impegni a valutare l'opportunità di dotare le Regioni degli strumenti finanziari necessari alla prosecuzione dei percorsi sperimentali d'istruzione e formazione professionale finalizzati anche all'assolvimento dell'obbligo scolastico.

che si riferisce ancora una volta al tentativo di dare soluzione interpretativa alle norme che regolamentano l'applicazione dell'ICI sui fabbricati rurali. Questo emendamento, di fatto, consente di porre fine a una serie di potenziali e reali contenziosi, che sono in atto e che continuano ad

come rurali; essi, nella prassi applicativa, diventano oggetto di imposta solo nel momento in cui si modificano le condizioni soggettive o oggettive del proprietario, quando viene a perdere il requisito della ruralità. Tra le diverse norme che si sono succedute, quella relativa all'iscrizione al catasto nonostante gli interventi ripetuti dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia del territorio, che hanno affermato che lo scopo della registrazione al catasto fosse esclusivamente finalizzato al censimento di tali unità immobiliari, senza che ciò comportasse effetti dal punto di vista fiscale - ha ingenerato una serie di interpretazioni della giurisprudenza, che ha dato e continua a dar luogo a contenziosi tra i Comuni e i proprietari dei fabbricati dotati dei requisiti della ruralità. L'emendamento vuole quindi fare chiarezza interpretativa, ribadendo le esenzioni ai fini fiscali afferenti ai fabbricati rurali purché vengano rispettati tutti i requisiti previsti dalle leggi. visto l'approssimarsi della scadenza di dicembre per il versamento del saldo ICI, nonostante ci sia un impegno già preso dal Governo ad emettere un provvedimento che ponga fine a tali contenziosi,

in quanto fino ad oggi le costruzioni rurali sono state esentate dall'ICI.

nell'attuale congiuntura economica, a facilitare Regioni ed enti locali, piuttosto che a comprimerli, nella gestione dei loro debiti finanziari. Non appare logico, infatti, né conveniente per tali enti sottoscrivere un prestito obbligazionario in forma fissa, per poi trasformarlo di fatto in un prestito obbligazionario ammortizzato a cui si associano spesso costi impliciti e di gestione. Appare altresì opportuno prevedere un obbligo di sottoscrivere strumenti finanziari solo se necessari alla riduzione del costo finale del debito sottoscritto e ad evitare che gli enti siano esposti a rischi di mercato, ancorché comprovati dai fatti degli ultimi tempi. Chiedo quindi di rivedere la normativa in materia, al fine di prevedere per Regioni ed enti locali la possibilità di rinegoziare o modificare i contratti aventi ad oggetto l'emissione di prestiti obbligazionari con rimborso del capitale a scadenza in forma fissa, i cosiddetti *bullet*, trasformando l'emissione obbligazionaria in forma ammortizzata, intendendosi risolti i cosiddetti contratti di *amortizing swap* o i *sinking funds*, in alternativa associati. In secondo luogo, con riferimento a posizioni di indebitamento a tasso fisso, prevedere il divieto per gli enti in questione di concludere operazioni di copertura in strumenti derivati, quantunque ai fini di ristrutturazione del debito, nonché di stipulare contratti derivati legati ai rischi di credito, laddove i medesimi comportino un'assunzione anziché un trasferimento di detti rischi.

Il retropensiero di questa norma sulla finanza pubblica porta a prevedere una centralizzazione della trattativa di tutta questa partita, che toglierebbe agli enti locali e agli enti territoriali la possibilità e l'autonomia di rinegoziare oggi le loro posizioni visto che quando hanno sottoscritto quei prodotti evidentemente non erano a conoscenza di tutto quel sottostante che poi abbiamo tristemente scoperto.

pertinenti agli interessi del Paese, ma la procedura che si è scelta per questa legge finanziaria e vi sarà certamente la possibilità di approfondire gli argomenti rappresentati dai vari emendamenti nei collegati o nei disegni di legge di merito specifico.

sotto un duplice profilo. Innanzi tutto, vi sono emendamenti di carattere ordinamentale e, come tali, pur avendo un valore intrinseco, non trovano sede nel disegno di legge finanziaria che - come noto - deve regolamentare esclusivamente questioni di carattere finanziario.

serve a finanziare l'attività dell'amministrazione; in essa, tra l'altro, sono presenti spese non solo per il funzionamento, ma anche per il pagamento del relativo personale. Sotto questo profilo, pertanto, utilizzare a copertura la tabella C significa sostanzialmente

pongono interessanti questioni in materia fiscale, che però postulerebbero la necessità di avere risorse più cospicue; questioni relative al finanziamento per il terremoto nel Belice, ma temo che si tratti di temi

da ultimo, un tema molto rilevante sollevato dal senatore Marino relativamente ai meccanismi di selezione per i ricercatori. Meccanismi per i quali,

NARDO *(IdV)*. Signora Presidente, onorevoli colleghi, è di questi giorni la notizia dell'ennesima emergenza alimentare. Sono state bloccate nel nostro Paese dai Carabinieri del nucleo antisofisticazione oltre 40 lotti di carni suine provenienti dall'Irlanda, contaminate da diossina in seguito all'uso, da parte dei coltivatori irlandesi, di mangimi inquinati da oli industriali. Sembrerebbe che gli stessi mangimi contaminati da diossina siano stati usati anche per gli allevamenti bovini. Chiedo che il Ministro competente venga urgentemente in Aula a riferire in merito alle citate notizie di stampa, che hanno creato un certo allarme tra i consumatori italiani, al fine di fornire corrette e dettagliate informazioni sui fatti richiamati,

nuovamente erogate le pensioni a coloro che, avendo usufruito dei benefici della legge sull'amianto, erano a qualche titolo coinvolti nelle inchieste della magistratura, senza però ricevere, per

altre a partire da dicembre. Dato che la pensione è l'elemento di sostentamento per queste persone, il problema è drammatico e rischia di diventarlo ancor di più. Il Ministro mi ha detto oggi che dovrebbe essere stata trasmessa ieri all'INPS la circolare che

ha detto che era disponibile ad una risposta scritta. Tradotto, ciò significa che, non essendoci contraddittorio, l'unica reazione che può avere colui che ha sottoscritto l'interrogazione è di presentarne una nuova in risposta

il Governo ancora una volta va in Abruzzo a dire delle cose, mentre in Aula, nelle sedi parlamentari, non fa il proprio dovere; ma, soprattutto - lo dico a lei in rappresentanza dell'intera Presidenza